che cortesemente la Presidenza mi abbia fatto sapere che era stato rivolto un sollecito al ministro Chiti, relativamente ad un'interrogazione sul piano scorte della Polizia di Stato.

In data 29 settembre 2006, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della solidarietà sociale:* «Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261,

*relatore*. Signor Presidente, in primo luogo, vorrei avanzare un'osservazione che riguarda i tempi della discussione e i caratteri dei due documenti al nostro esame;

È inutile che io indugi nel mettere in evidenza le difficoltà che derivano da questo stato di cose: la decisione di bilancio per il futuro interviene quando esso si è già trasformato pressoché totalmente in presente e, addirittura, in passato. Soprattutto, la decisione di bilancio per il futuro non può affondare radici sufficientemente solide nella resa dei conti dell'anno immediatamente precedente. Certo, i nostri uffici amministrativi ci consentono di avere cognizione anche dei dati di consuntivo 2005, ma non credo che questa conoscenza possa mettere rimedio ad un così grave ritardo della decisione. In proposito, tuttavia, si preannunciano novità positive: dal prossimo anno, grazie al nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione potrà essere elaborato, discusso ed approvato entro febbraio. Sempre dal prossimo esercizio, il conto consuntivo sarà quello dell'anno immediatamente precedente. È invece destinato a perdurare - signor Presidente, qui c'è un primo problema che vorrei segnalarle - il limite relativo alla natura del bilancio del Senato: il nuovo Regolamento contabile conferma, infatti, che continuerà ad essere solo un bilancio di cassa. Continuerà pertanto a sfuggirci - a causa della mancanza di un bilancio di competenza - il carattere prospettico delle decisioni di spesa e dei relativi oneri che via via il Senato assume, quando queste ultime, cioè le decisioni di spesa, siano destinate a determinare significative conseguenze nel tempo. Il comma 6 dell'articolo 2 del nuovo Regolamento contabile che prevede che il bilancio formulato in termini finanziari di cassa sia corredato da un allegato redatto in termini di competenza - è un passo avanti, ma non appare in grado di superare questo limite: sia perché l'allegato in questione è presentato ai soli fini di tipo cognitivo (non è oggetto della decisione di bilancio), sia perché il suo contenuto (contratti pluriennali e ammontare dei residui passivi) non è affatto esaustivo di ciò che troverebbe allocazione in un bilancio di competenza. Naturalmente, la presentazione di questo allegato costituisce un passo avanti, ma - ripeto - non è quello determinante. Per rendere più significativo questo passo avanti, il Senato - è la proposta che avanzo ai senatori Questori - potrebbe impegnare questi ultimi a disporre che, nell'allegato in questione, che, nell'allegato in questione, vengano contenute ulteriori informazioni, rispetto a quelle richiamate dall'articolo 2, comma 6, sulle tendenze pluriennali dei costi. Non sembrino queste, signor Presidente, questioni di mera tecnica contabile, sostanzialmente ininfluenti sulla decisione di bilancio vera e propria. Un esempio basterà per tutti, e certo la sua esperienza passata le consentirà di cogliere bene il punto: il Senato è sede di gestione di un sistema previdenziale, autonomamente regolato. Ogni decisione in questo campo - non importa se riferita ad un intervento sul sistema degli assegni vitalizi degli ex senatori o dei lavoratori dipendenti del Senato - non può e non deve essere assunta e valutata per gli effetti finanziari che determina negli anni immediatamente successivi, ma per la sostenibilità di medio e lungo periodo. Ciò che, per definizione, un bilancio dal respiro corto e cortissimo come quello formulato in termini finanziari di cassa non può fare. È appena il caso di ricordare, signor Presidente, che ancora oggi nel nostro Paese ci troviamo a fare i conti con le conseguenze di decisioni, in campo previdenziale, che furono assunte allora tanti anni fa - con valutazioni degli oneri limitate ai due o tre anni successivi al momento della decisione. Allo stesso modo, il carattere del bilancio di cassa non sembra idoneo a dar conto delle ragioni strutturali che presiedono alla decisione di impinguare i fondi di riserva. Perché impinguare i fondi di riserva in assenza di una visione prospettica di ciò che accadrà nei prossimi anni e in rapporto a ciò che è accaduto nel passato? Ancora: sulla base di un bilancio di cassa appare più problematico un rigoroso governo dell'evoluzione dei fondamentali aggregati di spesa (ad esempio, la retribuzione del personale),

integri l'allegato previsto dal comma 6 dell'articolo 2 dello stesso agendo come se si dovesse lavorare alla predisposizione di un bilancio di competenza. Vengo ora ad alcune considerazioni di merito sullo specifico progetto di bilancio al nostro esame. Lo faccio tenendo conto delle principali osservazioni emerse nel corso della riunione dei Presidenti delle Commissioni permanenti tenutasi nei giorni scorsi. In primo luogo, si segnala una significativa crescita della spesa per il personale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato (+ 7,1 per cento rispetto al 2005). Depurata la maggiore spesa dagli oneri derivanti da nuove assunzioni, l'incremento degli oneri per incrementi retributivi è pari a 8.500.000 euro, anche se resta più interessante il riferimento alle percentuali, che consente di comprendere meglio. In percentuale, l'incremento complessivo

Una dinamica, come si vede, ben al di sopra del tasso di inflazione programmata e tale da sollecitare, nel prossimo futuro, una più attenta verifica delle compatibilità finanziarie in sede di contrattazione. Sempre con riferimento alla spesa per il personale, va segnalata l'esigenza di superare un'evidente anomalia che si viene aggravando di anno in anno: tutti i dipendenti del Senato assunti dopo il 1998 non conoscono quale sia il loro trattamento previdenziale. Al contempo, ovviamente, il Senato non conosce l'evoluzione del debito pensionistico che si viene accumulando nei confronti di questa parte dei suoi dipendenti. A questa situazione si è giunti perché, nella fase successiva all'approvazione della riforma previdenziale del 1995 (la cosiddetta legge Dini), il Senato ha proceduto ad una revisione delle regole del sistema previdenziale dei lavoratori allora dipendenti, impegnandosi impegnandosi il Consiglio di Presidenza sin da allora a fissare regole nuove ma non determinate per coloro che fossero assunti dal 1998 in poi. Le nuove regole, da allora, non sono state fissate. Appare, quindi, indispensabile che si provveda immediatamente a porre fine a questo stato di incertezza, grave sia per le attese che suscita (è del tutto ovvio che in assenza di una deliberazione positiva tutti coloro che sono stati assunti dopo il 1998 sono ampiamente autorizzati ad attendersi che il loro sistema previdenziale sia uguale a quello dei lavoratori che già nel 1998 prestavano la loro attività presso il Senato), per l'alea cui espone l'equilibrio finanziario di lungo periodo del bilancio. In assenza di una decisione positiva si potrebbe giungere addirittura a decisioni che espongono ulteriormente il bilancio del Senato da questo punto di vista.

Nella Relazione sullo stato dell'Amministrazione (2006) si legge che «l'obiettivo primario è quello di garantire ai singoli senatori e agli organismi parlamentari (...) condizioni efficaci per il pieno e migliore svolgimento dell'attività parlamentare». parlamentare». L'esame del bilancio conduce ad una verifica positiva circa la capacità delle scelte allocative, compiute dal bilancio stesso, di conseguire questo fondamentale obiettivo, naturalmente in termini di giudizio generale. Va tuttavia segnalato che l'evoluzione di alcuni capitoli di spesa (nella relazione scritta faccio puntualmente riferimento ai capitoli) sembra testimoniare di un progressivo concentrarsi dell'attenzione vorrei dire aggiuntiva in termini di risorse, cioè della scelta di allocare risorse aggiuntive - verso attività,come le pubblicazioni, l'archivio storico e così via, rivolte all'iniziativa "esterna" del Senato (cioè del Senato verso l'esterno), piuttosto che a migliorare le *performance* del Senato sul fulcro della sua attività (la legislazione e l'attività di sindacato sull'attività del Governo). La dinamica della spesa in alcuni settori di attività "esterne" (più 100 per cento in cinque anni), certamente derivante dalla priorità riconosciuta a questo tipo di interventi (cito, per tutti, il caso dell'Archivio storico), suggerisce ora di provvedere ad un riequilibrio, signor Presidente, programmaticamente concentrato su quello che -chiedendo perdono ai costituzionalisti - chiamerò il *core business* dell'attività del Senato, cioè la nostra attività fondamentale. In proposito, la riunione dei Presidenti delle Commissioni permanenti ha fatto emergere due linee prioritarie di intervento, che io richiamo anche con qualche osservazione aggiuntiva rispetto alla relazione scritta.

o previste per l'immediato futuro a questo scopo, mi consentono di evitare una specifica elencazione degli interventi suggeriti dai Presidenti, alcuni dei quali considerati dai Presidenti stessi assolutamente urgenti in questo campo. La seconda, di più complessa attuazione, riguarda le attività di documentazione, ricerca e analisi, svolte dai Servizi del Senato e poste alla base dell'attività legislativa dei singoli senatori e del Senato nel suo complesso.

che ciascuna delle due Camere si doti, in perfetta autonomia rispetto all'altra, dei servizi di immediato supporto all'attività legislativa e di sindacato, altrettanto, signor Presidente, non può dirsi dei servizi di analisi e di documentazione

impongono scelte orientate al principio della intercameralità. Chiedo perché vi sono due biblioteche e non la biblioteca del Parlamento. Tra l'altro, a questo proposito, l'adozione molto opportuna di metodi e di strumenti di catalogazione identici tra Biblioteca della Camera e Biblioteca del Senato e la perfetta contiguità fisica delle attuali due Biblioteche sembrano rendere possibile, se non l'immediata unificazione, certamente la totale integrazione dal punto di vista dei fruitori delle due Biblioteche

non credo di proporle un obiettivo troppo ambizioso se le dico che forse nel 2007 quella porta si potrebbe aprire. Chiedo anche perché vi sono due Servizi del bilancio e non il Servizio del bilancio del Parlamento. Sarebbero pertanto opportune iniziative volte a coordinare da subito le attività di questi Servizi, con l'esplicito obiettivo di giungere in breve tempo a realizzare vere e proprie operazioni di unificazione. L'allargamento dell'area di intercameralità, in sostanza, consentirebbe di realizzare risparmi e di migliorare ulteriormente le prestazioni del Parlamento nel suo complesso. A questo punto, signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sul ruolo del Parlamento per assicurare un bene pubblico fondamentale, la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici italiani, oggi non assicurato in quantità e qualità sufficiente. Se un Paese con un debito pubblico come il nostro non ha sufficiente credibilità, quel Paese rischia sul versante economicamente rilevantissimo del merito di credito. Ora, la Corte dei conti, nell'ultima audizione sul DPEF, ha affermato esplicitamente:

tutta la decisione di bilancio è sottoposta a un rischio molto serio. Il Fondo monetario internazionale ha scritto nell'ultimo *outlook* sull'Italia che i conti pubblici italiani sono opachi. Questo è un problema aperto al quale la politica italiana deve dare una risposta. C'è chi ha sostenuto che questa risposta dovrebbe essere individuata nella costruzione di un'autorità fuori dal circuito Governo‑Parlamento e in particolare fuori dall'attività parlamentare. Personalmente, sono decisamente contrario a questa soluzione. Il modello di Governo italiano è un modello di Governo parlamentare, la trasparenza dei conti pubblici deve essere garantita da servizi di analisi di autorevolissimo livello assicurati dal Parlamento, ma si può seriamente sostenere, signor Presidente, che la Camera per sé o il Senato per sé siano in grado di offrire una risposta adeguata a questa esigenza questa esigenza primaria del Paese? Su questo punto nutro molti dubbi e penso che una scelta per il coordinamento e l'integrazione immediata dei due Servizi del bilancio per arrivare poi rapidamente, nel corso di questa legislatura, alla loro unificazione loro unificazione offrirebbe al Paese nel suo complesso una risposta di qualità a una domanda che altrimenti rischia di avere risposte alternative e di ulteriore dequalificazione. Infine, un cenno al tema dell'utilizzo degli spazi fisici. Mentre si sta uscendo molto rapidamente - e bisogna elogiare la struttura che si è occupata di questo intervento dalla situazione di emergenza determinata dalla ristrutturazione dei locali dell'ex Hotel Bologna, appare ragionevole ispirare la riallocazione delle diverse attività nelle diverse sedi a un principio di carattere generale:

Tutto ciò che serve al Senato per amministrare se stesso e sviluppare iniziative esterne può essere utilmente allocato nelle altre sedi a disposizione, ponendosi quindi anche per il Senato, signor Presidente, un problema che si pone per tutta la pubblica amministrazione italiana. La pubblica amministrazione italiana ha una caratteristica negativa, a paragone con quella di altri Paesi: impiega una quantità percentualmente più elevata di risorse per amministrare se stessa in rapporto alle risorse impiegate per produrre beni e servizi. dobbiamo, a mio avviso, operare una rivisitazione del bilancio - non è compito mio, naturalmente, ma dei senatori Questori e del Consiglio di Presidenza - alla luce di questo principio generale: meno risorse per governare noi stessi, più risorse per produrre

Questore*. Signor Presidente, colleghi, intervenendo in apertura di questo dibattito, per integrare le relazioni che accompagnano i documenti di bilancio oggi al vostro esame, anche a nome dei colleghi questori Thaler e Comincioli, desidero innanzitutto indirizzare all'intera Assemblea un doveroso saluto, rivolto in particolar modo al presidente Marini e ai senatori presenti, che ringrazio già fin d'ora per il prezioso contributo di approfondimento che vorranno portare alla discussione. Il nostro saluto va anche al Segretario generale, ai vertici dell'Amministrazione ed a tutto il personale che con noi collabora quotidianamente, mettendo a disposizione dell'attività parlamentare e dei senatori un patrimonio di professionalità e di dedizione di cui credo noi tutti dovremmo andare orgogliosi. È inevitabile, e dunque consuetudine, che nell'anno di passaggio da una legislatura all'altra sia la nuova Assemblea ad approvare il bilancio predisposto e deliberato rispettivamente dal Collegio dei senatori Questori e dal Consiglio di presidenza della legislatura uscente. Peraltro, diamo atto agli organi collegiali della precedente legislatura della sollecita approvazione dello strumento di bilancio, il che, nel passaggio particolarmente delicato e complesso da una legislatura all'altra, ha consentito certezza di risorse finanziarie e continuità alla concreta gestione amministrativa. Il Consiglio di Presidenza in carica, nella riunione del 27 luglio, prima della pausa estiva, ha preso atto dei documenti di bilancio deliberati sin dal 9 febbraio scorso, mentre il 20 dello scorso mese di settembre gli stessi atti, prima della discussione odierna in Assemblea, sono stati oggetto di esame da parte dei Presidenti delle Commissioni permanenti, lo ricordava il collega Morando, come previsto dall'articolo 165 del Regolamento del Senato. Il Collegio dei Questori, non lo nascondo, avrebbe voluto completare questi ultimi adempimenti prima della pausa estiva, ma non è stato possibile in ragione dell'intensa attività parlamentare che ha impegnato l'Assemblea, le Commissioni e lo stesso Consiglio di Presidenza nelle ultime settimane dello scorso mese di luglio. Per tale motivo, al pari di quanto sovente è accaduto negli anni in cui si tengono le elezioni politiche, la discussione odierna sul bilancio interno avviene quando sono ormai trascorsi oltre i due terzi e quindi pressoché in prossimità della chiusura dell'anno finanziario di riferimento. A tale proposito, il Collegio dei senatori Questori in questa sede assume l'impegno, per quanto di propria competenza, affinché negli anni futuri la discussione sul bilancio preventivo e sul rendiconto giunga all'attenzione dell'Assemblea nei termini più ravvicinati, a ridosso della deliberazione da parte del Consiglio di Presidenza prevista dal Regolamento di amministrazione e contabilità entro il termine del 28 febbraio. Il Collegio dei Questori, preso atto del progetto di bilancio interno a suo tempo deliberato, si è fatto carico nel corso di questi primi mesi di mandato di dare seguito alla linea progettuale ivi contenuta, anche perché convinto, supportato in questo dall'indirizzo espresso dal Consiglio di Presidenza nella citata riunione del 27 luglio scorso, dell'obiettivo strategico e assolutamente prioritario di portare a compimento gli interventi finalizzati a migliorare le condizioni per l'attività parlamentare, realizzando finalmente l'obiettivo di mettere a disposizione di ogni senatore, dei Gruppi parlamentari e degli uffici del Senato condizioni logistiche e strutturali adeguate al ruolo, al prestigio ed alle funzioni del Senato della Repubblica. A tale proposito, non possiamo che salutare positivamente il rispetto dei tempi di consegna dei lavori di adeguamento dell'ex Hotel Bologna, che da questo punto di vista inizia a restituire alla disponibilità del Senato e della sua funzionalità una rilevante ed importante struttura del patrimonio immobiliare. Per i contenuti e le analisi di dettaglio dei documenti di bilancio al vostro esame, mi rimetto alle ampie relazioni di accompagnamento. In questa sede mi limiterò, invece, a qualche essenziale considerazione su due soli profili del dibattito. Mi riferisco, da una parte, alle questioni sollevate in ordine ai costi della politica, e in particolare alla quantità di risorse destinate al funzionamento delle istituzioni parlamentari; dall'altra, alle istanze poste dalla relazione del presidente Morando rafforzate poc'anzi dal suo intervento - cui va il mio personale ringraziamento anche per aver evidenziato con estrema puntualità le problematiche emerse nel corso della già richiamata riunione dei Presidenti delle Commissioni permanenti. Una prima doverosa riflessione merita la *vexata quaestio* della misura della dotazione ordinaria prevista nel bilancio dello Stato a favore del Senato della Repubblica.

assunta dal Consiglio di Presidenza della precedente legislatura e pienamente condivisa dal Consiglio di Presidenza e dal Collegio dei senatori Questori neoeletti, di un taglio significativo alle previsioni originariamente formulate per gli esercizi 2006, 2007 e 2008, per cui le rispettive dotazioni ordinarie sono state ridotte da 501 a 487 milioni di euro, da 526 a 503 milioni di euro e da 552 a 519 milioni di euro. Il Senato ha assunto in piena autonomia tali decisioni, pur nell'ambito di un indirizzo coordinato con gli altri organi costituzionali e, sempre in tale ottica di coordinamento, anche nei prossimi anni si potrà considerare la possibilità di ulteriori possibili riduzioni di spesa, fatte salve le inderogabili esigenze di funzionamento di questa amministrazione. Ma non può e non deve sfuggire la circostanza che tale riduzione complessiva nel triennio è di ben 70 milioni di euro, per cento della richiesta originaria e addirittura superiore, in valore assoluto, di oltre un milione di euro rispetto all'analoga riduzione operata presso l'altro ramo del Parlamento. Tale riduzione rappresenta un contributo non indifferente del Senato alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, prospettate ancora oggi anche sugli organi di stampa. La cifra di 24 milioni di euro rappresentano un minor onere di bilancio, conseguente alla riduzione del 10 per cento operata sulle indennità dei senatori e sui trattamenti vitalizi. 46 milioni di euro si riferisce direttamente alle economie di spesa che il Senato autonomamente si è impegnato a realizzare nel triennio 2006‑2008, incidendo sulla struttura finanziaria del bilancio stesso. posti da un così rilevante taglio di risorse finanziarie, ancor più condizionante se considerato alla luce del carattere obbligatorio di oltre l'80 per cento (quindi, per definizione, insopprimibile), ha richiesto un'attenta definizione delle poste di bilancio, allo scopo di assicurare adeguata copertura finanziaria alle fondamentali esigenze di ordinario funzionamento dell'istituzione e ai rilevanti principali interventi a carattere straordinario già avviati, soprattutto nei settori immobiliare, delle infrastrutture informatiche e della sicurezza. La consistenza stessa degli stanziamenti iscritti sui capitoli dei fondi di riserva per le spese impreviste è espressione del rigore, ma anche del ragionevole equilibrio che caratterizzano il progetto di bilancio per il 2006. Essi hanno garantito adeguata copertura finanziaria anche ad alcuni provvedimenti, adottati su proposta dei senatori Questori dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 1º giugno scorso. Riguardo alle questioni poste dalla relazione del presidente Morando, poc'anzi egregiamente richiamate, mi limiterò ad approfondire nel merito solo quelle che riguardano più direttamente i profili del bilancio. Per il resto, si possono condividere le considerazioni svolte nell'ultima parte dell'accennata relazione, in ordine alla prospettata esigenza di dare impulso ad iniziative che coinvolgano, ovviamente, anche la Camera dei deputati, volte a razionalizzare, ai fini di una migliore efficacia, alcune strutture attualmente esistenti, che consentirebbero di perseguire in coordinamento obiettivi di ottimizzazione dell'uso delle risorse, di rafforzamento in termini di efficienza e di prestigio, nonché una più adeguata visibilità dell'istituzione Parlamento nel suo complesso. Nella sua relazione, il presidente Morando evidenzia l'opportunità di affiancare all'attuale bilancio finanziario, espresso in termini di cassa, un bilancio formulato in termini di competenza finanziaria. Torna così, in questa sede, un dibattito non non nuovo, che ha sempre appassionato gli esperti di contabilità pubblica. Quello che si può affermare è che sull'orientamento assunto dalla Commissione di esperti presieduta dal professor Roversi Monaco, che ha elaborato il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, circa il mantenimento del solo bilancio finanziario di cassa hanno certamente influito il dibattito e le regolamentazioni che vanno accompagnando le riforme dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. Si va, infatti, gradualmente affermando la tendenza ad un sistema di contabilità che vede il progressivo abbandono del bilancio di competenza giuridico-finanziaria, quale fin qui conosciuto, per l'adozione in sua vece di un bilancio di competenza economica che, affiancato da un documento di cassa, offra una migliore informazione circa la congruità tra risorse assegnate e risultati amministrativi raggiunti. Peraltro, il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità l'adozione di strumenti e procedure finalizzate ad informare espressamente la gestione del bilancio e l'azione amministrativa al principio della programmazione; l'esame del bilancio di previsione congiuntamente al rendiconto dell'anno immediatamente precedente; infine, l'obbligo di presentare a corredo del documento di bilancio gli allegati dei dati in termini di competenza cui si faceva riferimento cioè quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 2 del nuovo Regolamento - che indichino gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione di contratti pluriennali in corso di validità e l'ammontare presunto dei residui passivi. Tali innovazioni, ulteriormente rafforzabili con il suggerimento poc'anzi avanzato dal presidente Morando, possono essere considerate una risposta positiva a molte delle esigenze poste nel corso di queste riflessioni. Debbo aggiungere che lo stesso Regolamento di amministrazione e contabilità com'è stato ben sottolineato dal Consiglio di Presidenza all'atto del suo esame - è soggetto ad ulteriori modifiche alla luce di una prima attuazione dei suoi contenuti. Saranno, pertanto, seguiti con particolare attenzione tutti gli aspetti funzionali e operativi connessi all'applicazione del nuovo strumento regolamentare, che diventerà pienamente operativo dal prossimo anno, allo scopo di verificarne la piena rispondenza agli obiettivi che ci siamo posti, sollevati anche dal presidente Morando, di una più adeguata e trasparente gestione del nostro bilancio. In ogni caso, le sollecitazioni rappresentate nella relazione del collega Morando saranno oggetto di ulteriori approfondimenti, volti a considerare la possibilità di adottare anche in Senato schemi di contabilità economica che tengano conto delle evoluzioni ed anche delle problematiche che si vanno evidenziando con riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche, che non sono certamente estranee - né possono esserlo - all'amministrazione del Senato. Per altro verso, occorre rilevare che alcune delle esigenze informative, quali quelle relative alla spesa pensionistica, non possono essere soddisfatte attraverso i dati di bilancio comunque costruiti, ma devono essere oggetto di specifiche indagini prospettiche. Si tratta di informazioni di carattere necessariamente aggiuntivo rispetto ai bilanci che possono, insieme ad altre, quali i citati andamenti della spesa per il personale, gli investimenti immobiliari e programmi di informatizzazione, trovare riscontro in specifici documenti di programmazione economica e finanziaria. In tal senso, il Consiglio di Presidenza ha già disposto specifiche indagini di carattere attuariale anche in ordine al sistema pensionistico vigente per i dipendenti del Senato della Repubblica, incluso il riferimento alla necessità di prevedere, e di provvedere finalmente, ad un preciso regime previdenziale per coloro i quali sono stati assunti dal 1° gennaio 1998, colmando in tale modo una lacuna normativa che ormai perdura da troppo tempo e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale hanno fortemente sollecitato affinché venga colmata.

criteri più rigorosi ai fini del collocamento a riposo e, dall'altro, dall'esigenza di evitare il diffondersi di inappropriati allarmismi tra il personale circa i diritti acquisiti e le posizioni già maturate. Interventi di modifica al sistema vigente, anche mediante la previsione di apposite norme transitorie, credo dovranno tenere conto di questa pregiudiziale esigenza. Non posso nascondere che, nel corso delle ultime settimane, abbiamo avuto una richiesta di quiescenza di collocamento in pensione assolutamente spropositata rispetto alla media annuale vigente qui al Senato, dovuta probabilmente al diffondersi di paure e preoccupazioni che ritengo assolutamente infondate e spero che, anche alla luce dell'odierno dibattito e di questa discussione, possano rientrare. La relazione del presidente Morando evidenzia, inoltre, alcune preoccupazioni in ordine all'andamento della spesa complessiva di questa amministrazione; al di là delle opinioni più estreme e meno informate che nel tempo hanno suggerito la necessità di un blocco della spesa del Senato, un confronto che possa apparire nel contempo serio e significativo dovrebbe considerare l'andamento della spesa corrente del Senato rispetto all'andamento della spesa corrente dello Stato, al netto degli interessi. Possono essere d'ausilio, a tal fine, le appendici statistiche contenute nell'ultima relazione della Corte dei conti sul rendiconto dello Stato per l'anno 2005 e che considerano il periodo 1997-2005. La spesa corrente dello Stato, ripeto, al netto degli interessi, registra nel periodo 1997-2005 un aumento del 75 per cento, in termini di pagamenti, mentre la spesa corrente del Senato evidenzia, nel medesimo periodo, un aumento del 64 Valutazioni analoghe possono essere espresse con riferimento, in particolare, alla spesa per le retribuzioni del personale di ruolo ed a contratto a tempo indeterminato. Considerando, come suggeriscono le stesse analisi condotte dalla Corte dei conti, l'andamento della retribuzione *pro capite*, il dato significativo espresso dall'ultimo quinquennio presenta, nel caso delle pubbliche amministrazioni, un tasso di aumento del 24,01 per cento, a fronte di un incremento, nello stesso periodo di riferimento, del 23,22 per cento della retribuzione *pro capite* dei dipendenti del Senato. Ad onor del vero, va anche ricordato, sempre sulla questione delle retribuzioni dei dipendenti, che il loro andamento risente anche degli effetti economici previsti da uno specifico accordo contrattuale in materia di incremento di produttività, sulla base di maggiori prestazioni di servizio (il ripristino delle 40 ore settimanali, ad esempio, contro le 37,5) e la rinuncia ad alcune giornate di ferie in cambio di un incremento retributivo.

nei diversi piani, un certo numero di personale che svolga anche compiti di sicurezza. Per rispettare tali norme, abbiamo bisogno di una dotazione organica e di un monte ore di lavoro che, grazie a questo accordo, è stato possibile conseguire. Debbo anche dire che si tratta di un caso tratta di un caso probabilmente unico nella storia della contrattazione pubblica degli ultimi anni. Solo così si può spiegare lo scostamento dal 4,5 per cento, dato di crescita dei redditi da lavoro dipendente,

Infine, anche i dati, di cui alla tabella esposta a pagina 5 della relazione di accompagnamento al progetto di bilancio per il 2006, evidenziano l'impegno posto dal Senato, in questi anni di difficoltà della finanza pubblica, con l'obiettivo di ridurre negli anni la curva di incremento delle risorse complessive e, conseguentemente, della propria spesa. Naturalmente, tali dati nulla tolgono all'opportunità di misure di contenimento della spesa per il futuro e le decisioni di spesa del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori dovranno continuare ad essere coerenti con questo obiettivo anche nei prossimi anni. succitati dati riportano su un piano realistico e di correttezza alcune opinioni che sono state espresse in ordine a un incontrollato e abnorme aumento della spesa del Senato negli ultimi anni. Signor Presidente, colleghi, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, i senatori Questori ritengono che il progetto di bilancio di previsione per il 2006 risponda a quegli obiettivi di contenimento della spesa imposti dalla particolare situazione finanziaria del Paese e, sotto questo profilo, esso rappresenta per noi un solido punto di partenza, non certo di arrivo. Identici, rigorosi obiettivi dovranno essere perseguiti anche negli anni futuri e trovare compiuta espressione: tale è l'impegno dei senatori Questori a partire dal bilancio di previsione del prossimo anno. Infatti, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, a partire dal 2007 siamo chiamati a disegnare una nuova struttura espositiva del bilancio, più snella e più adeguata alle concrete esigenze della gestione, che risponda altresì a criteri di trasparenza e di migliore leggibilità. In quella sede ci ripromettiamo di intervenire, ovviamente, sulla definizione e sull'allocazione delle risorse, predisponendo un bilancio di previsione che evidenzi la coerenza del documento finanziario con i programmi che insieme al Consiglio di Presidenza si vorranno adottare, in ordine al perseguimento di obiettivi di sempre maggiore efficienza della macchina amministrativa interna al servizio dell'attività parlamentare e, comunque, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei già richiamati obiettivi di contenimento della spesa. Si tratta di traguardi che intendiamo conseguire, anche se nei prossimi mesi il loro pieno perseguimento richiederà, da parte di questo Collegio e della struttura amministrativa, un'attività particolarmente intensa. Ma, come si è già detto in precedenza, siamo determinati a sottoporre al Consiglio di Presidenza, nel rispetto del termine regolamentare del 28 febbraio prossimo, sia il progetto di bilancio per il 2007, sia il rendiconto del bilancio 2006, così come previsto dal nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità che in ciò ha portato una radicale innovazione rispetto alla disciplina in vigore. Riteniamo che l'esame dei documenti di bilancio nelle diverse sedi previste dall'*iter* procedurale - Consiglio di Presidenza, Conferenza dei Presidenti di Commissione e infine - possa costituire con il contributo di tutti un momento di confronto e di arricchimento per la vita e la gestione di questa istituzione. In definitiva, siamo convinti siano questi l'auspicio e l'obiettivo del nostro dibattito. In conclusione, chiedo all'Assemblea di approvare il progetto di bilancio per l'anno finanziario 2006 ed il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario

tratta, infatti, di una situazione di disagio che non è giusto mantenere. Una situazione di incertezza in questo campo è sempre portatrice di difficoltà e non è mai

soprattutto per l'impostazione del bilancio 2007, per rendere l'istituzione Senato sempre più efficiente e rispondente alla sua funzione.

Occorre riconoscere gli sforzi fatti per tenere il passo nel processo di informatizzazione, sia con gli strumenti informatici di cui i senatori hanno beneficiato che nelle reti infrastrutturali. Va riconosciuto che le decisioni del 2001 hanno consentito ai senatori di trovarsi in una condizione privilegiata rispetto alla Camera in termini di collegamento funzionale. Di questo ce ne eravamo fatti carico noi stessi. Oggi l'informazione viaggia sulla rete e ciò consente un maggior dialogo sia con gli elettori, anche in considerazione dei vasti collegi regionali, sia con i «mondi vitali». Dobbiamo allora rafforzare questi strumenti se vogliamo giungere a decisioni corrette, soprattutto nella piena consapevolezza degli effetti. In questa direzione, onorevole Questore, si muove l'ordine del giorno G4, presentato per il collegamento informatico con il Ministero dell'economia e delle finanze. Oggi quei dati, soprattutto quelli fiscali, sono indispensabili se vogliamo riequilibrare un rapporto Governo-Parlamento che si è alterato progressivamente e che va invece ricalibrato. La centralità parlamentare non può essere solo uno *slogan* da

avere la disponibilità dei dati fiscali significa confrontarsi in modo dialettico ed efficace e non subire il dominio di soggetti esterni. A tale riguardo, vorrei ricordare, onorevole Questore, onorevole Presidente, che nella scorsa legislatura affrontai in ogni sede - lo sottolineo - sia in Aula sia in Commissione, il problema del ritorno al pubblico della società SOGEI che, nella sciagurata privatizzazione di Telecom, era diventata di proprietà privata insieme a tutti quei dati sensibili dei contribuenti italiani che potevano essere nella disponibilità di taluni e anche di alcune trame oscure, come ha dimostrato la recentissima vicenda. Ed i fatti ci hanno dato ragione. Le vicende dei giorni scorsi hanno confermato l'attenzione e l'azione verso quei dati, che dovevano restare nell'ambito di una adeguata tutela pubblica, la cui salvaguardia passava per il mantenimento della proprietà. Un'altra questione, su cui riflettere, è quella dei costi della politica. fa molta demagogia in questi giorni, quasi una gara a presentare proposte estemporanee, che alimentano un distacco dell'opinione pubblica. Lo scorso anno, onorevole Presidente, fui unico a contrastare il ministro Tremonti rispetto al famoso taglio del 10 per cento delle indennità, ma non perché fossi contrario soltanto a titolo personale. No! Credo che su tale questione si debba procedere come si è fatto quest'anno, onorevole Questore, anche con forte economia di spesa, ma per autodisciplina e per autocontenimento: all'interno del volume delle risorse, cioè, lo stesso Senato e la stessa Camera devono poter decidere il *quantum* da poter contenere perché storicamente il bilancio appartiene al Parlamento. È il Parlamento che decide le risorse da spendere e non deve subire imposizioni. Non possiamo mettere in discussione questo principio storico anche perché gli sprechi non si annidano qui dentro, onorevole Questore. Nei giorni scorsi, leggevo di una Regione, definita il Circo Barnum,

è un livello di spesa che non si può abbassare, pena un peggioramento della qualità dei servizi e la qualità delle risorse umane, di grande professionalità, di cui oggi disponiamo, impegnate nello svolgimento di servizi visibili, ma anche di servizi invisibili, ma tutti di identica efficienza, rilevanza e responsabilità. e responsabilità. Dobbiamo stare attenti ad equiparare il Senato e coinvolgerlo nell'indistinto della pubblica amministrazione, come ha cercato di fare poco fa il senatore Morando. Credo sia un bene da salvaguardare senza demagogia. Quando si fa un parallelo tra l'incremento della spesa del Senato per il personale del 5,7

di produttività, che pure è stato realizzato attraverso una maggiore disponibilità al sacrificio e agli orari. C'è poi un problema strettamente collegato a quello delle indennità parlamentari: il problema delle incompatibilità. Viene da domandarsi se non siano superate quelle disposizioni che impediscono ad alcune categorie di dipendenti di svolgere la professione originaria, come i professori universitari, gli insegnanti, i medici pubblici, costretti all'aspettativa, a fronte di altri liberi professionisti, come avvocati, presentatori televisivi, giornalisti, che, al contrario, possono svolgere libere professioni senza preclusioni. Se questo è, significa che si determinano due categorie di parlamentari - quelli di serie A e quelli di serie B - e tutto ciò finisce per impoverire la qualità della rappresentanza, limitando perfino a ceti e categorie la possibilità di essere rappresentati in Parlamento. Questori queste osservazioni, confidando naturalmente nell'accoglimento degli ordini del giorno presentati e, soprattutto, nella predisposizione del progetto di bilancio 2007, affinché possano essere affrontate le questioni che diano il senso di un progetto di legislatura, superando le difficoltà contingenti, e quindi rispetto ad un orizzonte progettuale. Esprimo, pertanto, un giudizio positivo rispetto all'impostazione del bilancio, ma non posso non lumeggiare una questione sulla quale mi ero soffermato anche nell'Ufficio di Presidenza.

Proprio perché si tratta di una riforma di sistema, come quella del nuovo Regolamento, è bene precisare che sarebbe stato necessario affiancare i due sistemi contabili: al sistema di contabilità pubblico‑finanziaria, il sistema di contabilità economico‑analitica, al fine del monitoraggio più efficace, più efficiente e più economico dell'azione amministrativa e per il conseguente controllo di gestione. È mancato, infatti, onorevole Presidente e onorevole relatore, l'introduzione del controllo di gestione che è lo strumento guida ai fini della sana gestione amministrativa (tutto ciò in base alle direttive europee contemplate nel decreto legislativo n. Tale strumento avrebbe permesso la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione, elemento questo non realizzabile attraverso il mero controllo di di legittimità, ritenuto anacronistico e non sufficiente ai fini della sana gestione amministrativa. È stata però soppressa l'idea stessa, che avevo sostenuto, del controllo di gestione: ero e sono dell'idea di prevedere l'introduzione di questa rilevante innovazione e l'istituzione, appunto, delle unità di controllo, che sarebbe risultata di grande utilità ai fini del passaggio ad una logica di programmazione e controllo richiamata, anche questa, dal senatore Morando nella relazione. Ma, onorevole Morando,

Rafforzare l'istituzione parlamentare nel suo complesso significa rafforzare la democrazia nell'interesse non di ciascuno di noi, ma del Paese. Per tali ragioni, esprimo un giudizio positivo e il mio apprezzamento per le scelte operate, naturalmente auspicando che queste indicazioni, che mi sono permesso di sottolineare, possano trovare maggiore spazio nel progetto di bilancio 2007.

la problematica che pongo all'attenzione dell'Aula non vuole avere - lo preciso - un carattere moralistico, meno che mai sembrare una battaglia donchisciottesca. la problematica dei collaboratori parlamentari nella qualità di neosenatore. Nei primi mesi di presenza a Roma ho avuto modo di parlare con circa 30 giovani, diplomati, laureati, alcuni anche con un doppio titolo di laurea, che hanno svolto - mi hanno detto - alcuni per pochi anni, altri anche per un decennio e passa, la loro prestazione professionale sia per parlamentari della Camera e del Senato, sia per il raggruppamento di centro-destra e di centro‑sinistra. Bene, questi giovani - richiamo l'attenzione dei colleghi distratti, perché parlo non solo alla loro razionalità, ma anche alla loro coscienza - hanno confessato candidamente di non avere nessun anno di contribuzione previdenziale e assicurativa perché hanno sempre percepito tra i 500 e i 1.500 euro al mese, ma senza contribuzione, cioè al nero. Alcuni mi hanno anche precisato che, allorquando il proprio parlamentare di riferimento è divenuto membro del Governo oppure ha assunto incarichi qualificanti (quali Presidente di Commissione, Questore, Segretario, membro dell'Ufficio di Presidenza), si sono ritrovati ad avere il trattamento economico a carico dell'amministrazione e, come per magia, i loro stipendi, grazie alla benevolenza delle amministrazioni, si sono

in termini di giustizia per un lavoro nero che così ci è vicino e che invece in quest'Aula, così come nell'altro ramo del Parlamento, spesso con enfasi retorica - io aggiungerei, mi scuserete, anche con molta ipocrisia tanti stigmatizzano, avendo vicino a loro situazioni similari. Ma dicevo prima del carattere non moralistico della problematica che pongo, perché intendo difendere anche lo stesso parlamentare. Come amabilmente mi ha fatto scrivere il Ministro del lavoro dalla sua direttrice generale Lea Battistoni, c'è l'assenza di una qualificazione normativa; cioè, il parlamentare che vuole comportarsi - come è giusto - correttamente, ha difficoltà a trovare uno strumento normativo di riferimento chiaro e preciso. È vero che esistono i contratti a termine, è vero che esiste la possibilità di pagare le prestazioni quali prestazioni professionali su fattura; ma queste, colleghi, sono delle forzature, ricordiamocelo. Lo stesso INPS ha posto la questione; sono delle forzature, non è ammissibile. Il collaboratore parlamentare, infatti, svolge la sua attività munito di *badge* identificativo rilasciato dagli Uffici di questura dei due rami del Parlamento; accede agli spazi, ai palazzi di proprietà e/o di competenza (quando sono in locazione) dei due rami del Parlamento; utilizza, in una sorta di comodato gratuito, uffici, arredi, strumenti, reti insieme al proprio parlamentare, in un rapporto sì fiduciario, che tale è e tale deve rimanere, ma che certamente non può essere come accade in molti casi - strumentalizzato da un contratto a progetto solo ai fini di pagare minori oneri previdenziali e assicurativi. È molto scorretto ciò che accade. So che è quasi dalla nascita della Repubblica

bozze di disegni di legge o di interrogazioni parlamentari che poi il parlamentare completa, corregge o modifica secondo i suoi intendimenti.

«Mi corre l'obbligo di precisarle che il contributo per il supporto di attività e compiti degli onorevoli senatori connessi con lo svolgimento del mandato parlamentare, erogato mensilmente, non ha alcun vincolo di destinazione rispetto ad eventuali prestazioni lavorative rese da terzi o a possibili configurazioni contrattuali».

dal Senato, sia pure senza l'emissione di un formale cedolino, come forse sarebbe dovuto, quale indennità per le attività di supporto,

il presidente Marini, che ha una lunga e gloriosa militanza sindacale, ascoltasse direttamente questa mia segnalazione, perché probabilmente l'avrebbe

dei diritti che diventano privilegi piuttosto che alle necessità che rappresentano i veri diritti delle nuove generazioni. Spero, quindi, che il Collegio dei senatori Questori ed il Consiglio di Presidenza, al di là della mia modestissima proposta,

alle informazioni sui *badge* identificativi delle persone che entrano in Senato come collaboratori, scoprirebbero pochissime iscrizioni contributive. Questa non è cosa da Paese civile! Allora, mi auguro che il Collegio dei senatori Questori e il Consiglio di Presidenza sappiano svolgere un'indagine o meglio sappiano fare una segnalazione o una proposta seria, preferibilmente in modo coerente con l'altro ramo del Parlamento; piuttosto che pensare ad un'assunzione globale, dovrebbero identificare, entro un mese o due, una normativa specifica per i collaboratori parlamentari, la cui

e, in particolare, dal senatore Questore Nieddu, qui presente. Passo, quindi, ad illustrare molto rapidamente l'ordine del giorno G5. Il Consiglio di Presidenza ha approvato, con una

che tale decisione non abbia aspetti positivi sull'andamento dei lavori del Senato.

insegna che non vi è stato alcun miglioramento in questa direzione. Abbiamo altresì visto, nelle ultime votazioni, che, con un'Aula piena o quasi, come generalmente si verifica in particolare in questa legislatura, si individua molto bene la presenza o l'assenza dei senatori in occasione delle votazioni. Pertanto, non si avrebbe alcun beneficio dall'obbligo di stare in una determinata postazione per esprimere il proprio voto, viceversa, ci sarebbero diversi aspetti di scomodità e in diverse circostanze l'impossibilità di esprimere di esprimere il voto e di muoversi nell'ambito di quest'Aula, che è abbastanza piccola e raccolta per invitare a quella riflessione particolare alla quale il Senato dovrebbe essere particolarmente portato. Aggiungo un dettaglio molto materiale: alla Camera, dove da tempo c'è il posto fisso, le postazioni sono molto più ampie, cioè è possibile spostarsi senza che i colleghi della stessa fila debbano alzarsi; credo che chiunque sia stato deputato o semplicemente chiunque si sia seduto su un banco della Camera in occasione delle riunioni del Parlamento in seduta comune lo possa constatare.

però un vuoto informativo che a mio avviso il questore Nieddu dovrebbe colmare per dare chiarezza agli impegni che assumiamo in Aula: come

mi sembra più corretto, e forse anche più semplice, perché molto positivamente il Collegio ha già allegato

approvare nel Consiglio di Presidenza e in Assemblea il rendiconto per il 2005. Questo ci metterebbe immediatamente nelle condizioni di poter approvare a febbraio il rendiconto 2006 e la previsione 2007.

Se riuscissimo in tutta questa operazione, penso che faremmo opera meritoria, perché dare trasparenza ai documenti di bilancio, sia consuntivo che preventivo, è una delle cose più meritorie che si possano fare ed è anche un buon esempio. signor Presidente, si è aperto un dibattito questa mattina di un qualche interesse, anche perché se ne parla da tanto tempo, sull'utilità di fare il bilancio di cassa o il bilancio di competenza; è una bella discussione, personalmente propendo più per un bilancio di cassa, ma non sono alieno dal ritenere che vi siano ragioni anche dalla parte di chi sostiene l'utilità di un bilancio di competenza. Personalmente, credo che quest'anno il Collegio dei Questori e il Consiglio di presidenza abbiano adottato la soluzione migliore, quella di mantenere il bilancio di competenza, che dà una trasparenza e una visibilità immediate ed evita tanti problemi di gestione

che consentono all'Assemblea di avere un quadro abbastanza articolato, ma anche definito, degli impegni pluriennali. Comunque, la discussione è interessante, ho visto che anche il senatore questore Nieddu ha dedicato una certa attenzione al problema e secondo me è utile che si arrivi ad una conclusione definitiva, ma non propenderei per una soluzione *tout court* a favore del bilancio di competenza, personalmente ritengo che la soluzione adottata quest'anno sia quella più congeniale e conveniente per un'Assemblea elettiva. Del bilancio sottolineo un aspetto fortemente positivo, che noi assumiamo in continuità con la precedente gestione: la riduzione di ben 14 milioni di euro della dotazione annuale. È un fatto molto importante, rispetto al *trend* di spesa a favore del Senato, il trasferimento da parte del Governo di una quota ridotta di 14 milioni, mentre si svolge un'opera di risanamento e mentre abbiamo di fronte la necessità di ridurre la spesa pubblica; penso che il Senato dia un segnale di grandissima importanza.

Siccome siamo sempre portati alla cronaca per gli aspetti di maggiore spesa, penso sia doveroso che segnaliamo in maniera anche forte che questa volta dobbiamo passare alla cronaca perché

cioè, di risparmi che si ottengono sull'andamento della spesa corrente, rinviando di fatto i pagamenti all'anno successivo, ma di veri e propri risparmi di amministrazione.

completare i progetti avviati, arricchire le strutture immobiliari, potenziare i servizi informatici, irrobustire gli interventi per la sicurezza, qualificare sempre di più il nostro personale.

In primo luogo, suggerirei ai Questori, se possibile già quest'anno, altrimenti a partire dal prossimo, di aumentare il contributo per i Gruppi,

le consulenze esterne per il patrocinio del Senato. Personalmente ritengo che si debba provvedere attraverso l'avvocatura del Senato, affinché ci si doti in maniera strutturale di una difesa

parola in merito agli interventi in generale. Non ho presentato ordini del giorno perché ho piena fiducia che il Collegio dei senatori Questori terrà conto di tutte le osservazioni che i colleghi stanno svolgendo in questo dibattito.

In effetti, il senatore vive qui dentro dalla mattina alla sera per tre giorni e deve essere messo nella condizione di poter svolgere il proprio mandato al meglio. Questo mi pare debba essere l'obiettivo principale dei senatori

per gli aspetti logistici, invece, si può fare qualcosa di più. Vi sono situazioni che comportano perdite di tempo e disfunzioni; per non essere generico ne vorrei indicare alcune, pregando il senatore Questore Nieddu di dedicarvi attenzione.

palazzi) in maniera molto fastidiosa, anche perché è difficile districarsi in questi ambienti. Credo sia necessario, anzi indispensabile, istituire uno "Sportello unico",

a questo sportello unico diramare tutte le richieste e fornire successivamente le risposte ai senatori. Non è, però, corretto né efficiente che il senatore debba andare in giro per gli uffici del Palazzo a disbrigare le sue questioni. In secondo luogo, se un senatore desidera scrivere una lettera, preparare un intervento scritto, svolgere una qualsiasi attività nel Palazzo, soprattutto nei pressi dell'Aula, non può praticamente farlo. Non ci sono posti all'uopo attrezzati con scrittoi, fogli, buste, penne o telefoni: vi sono solo due sedie ed un tavolo, in un viavai continuo, nella stanza delle caselle. Eppure è una necessità per i senatori poter lavorare nei pressi dell'Aula, soprattutto per il disbrigo della posta o per la preparazione di un comunicato stampa. Ebbene, vi sono tre stanze tra l'Aula e il Transatlantico (la Sala della Firma, la Sala del Risorgimento e la Sala Marconi) che sono pressoché inutilizzate, se non come sale di passaggio o chiacchiericcio, con tavoli ornamentali al centro, senza sedie, senza scrittoi, senza fogli, senza buste, senza telefoni

(penso soprattutto al disbrigo della posta, alla preparazione degli interventi e ad un minimo di attività) che favorirebbero il disbrigo delle competenze l'utilizzazione della Sala Maccari. Se questa dev'essere una sala di lettura dei giornali e delle riviste, se deve servire per svolgere un qualche approfondimento,

che, adeguatamente adibita, anziché essere un vero e proprio corridoio, potrebbe avere un'utilizzazione di questo genere.

Se un senatore, nel corso della giornata, vuole ricevere una persona per un breve periodo o una delegazione per una riunione collegata ai lavori dell'Assemblea, praticamente non lo può fare. Questo perché nel Palazzo si possono incontrare le persone vicino all'ingresso, in un ambito angusto, senza nessuna riservatezza e, diciamo la verità, anche senza dignità per il senatore che riceve un ospite e per l'istituzione stessa. Deve essere trovato un qualche posto nel Palazzo dove il senatore possa ricevere un ospite dignitosamente. A me è venuta un'idea, ma ce ne possono essere tante altre: penso, ad esempio, all'atrio dell'ingresso di via della Dogana

di quello dove oggi, ahimè, avvengono questi incontri. Infine, Presidente, è stato affrontato il problema della comunicazione esterna. Navigare sul sito del Senato...

il passare del tempo, cambiano anche le opinioni; noi comunque rimaniamo favorevoli al provvedimento e quindi ci auguriamo che possa essere per l'attenzione i senatori Questori e l'Ufficio di Presidenza e soprattutto ringrazio tutti i dipendenti del Senato per la collaborazione che ci danno.

che si metta mano, e si risolva finalmente, la questione dei bagni perché, per quantità e qualità, soprattutto quelli riservati alle signore senatrici, sono veramente dei disservizi igienici più che servizi igienici.

emerga, assieme ad un giudizio positivo sulla proposta di bilancio che ci è stata presentata e di rendiconto 2004, anche una linea di intervento per il futuro che, del resto, in larga misura il senatore questore Nieddu ha già mostrato di voler far propria. Credo, quindi, di non dover aggiungere nulla, se non sollecitare i presentatori dei diversi ordini del giorno a considerare il fatto che in quegli ordini del giorno che hanno una ricaduta diretta su questioni che riguardano il Regolamento del Senato in senso stretto (e non il suo bilancio) non so con

o non ho un opinione precisa o, se ce l'ho, ce l'ho in quanto senatore, senza alcun riferimento ad un dibattito che si sia svolto in qualche sede.

fornire il loro contributo al nostro dibattito. In particolare, ringrazio il senatore Eufemi per aver richiamato, in un giudizio complessivamente positivo del nostro bilancio interno, l'impegno posto dai senatori Questori e dalle strutture amministrative per il raggiungimento degli obiettivi prioritari in ordine alla riqualificazione degli spazi, di dotare tutti i senatori di un ufficio adeguato al loro ruolo e alle funzioni del mandato parlamentare, ed al crescente miglioramento delle infrastrutture informatiche. Si terrà conto, in sede di prima applicazione del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, delle sue stimolanti riflessioni in ordine alla necessità di accompagnare l'azione programmatica della gestione di bilancio con adeguati strumenti e funzioni di controllo. Devo aggiungere che condivido, in modo particolare, la sottolineatura

una dinamica di gestione e di scelta politica che va verso la riduzione dei costi e il contenimento degli oneri. Passando agli ordini del giorno illustrati, il problema segnalato dal senatore Eufemi con l'ordine del giorno G4, è di estrema importanza e richiama delicate questioni di carattere politico-istituzionale, concernenti il rapporto tra Governo e Parlamento. In tal senso, la questione supera le competenze dei senatori Questori ed i limiti del bilancio interno, ma non vi è dubbio che esiste il problema di una conoscenza tempestiva e completa da parte del Parlamento degli andamenti delle entrate pubbliche, ai fini di una consapevole decisione politica. Infatti, con il decreto-legge n. 70 del 1988, fu prevista del 1988, fu prevista l'attivazione di un collegamento dei due rami del Parlamento al sistema informativo del Ministero delle finanze (ora dell'economia e delle finanze) gestito dalla SOGEI. Tale collegamento è stato attivato per la prima volta nel 1991. Per quanto concerne il Senato, esso è stato inizialmente attivato presso la Commissione finanze e tesoro per poi essere esteso anche agli uffici del Servizio del bilancio. Attualmente il collegamento si realizza attraverso Internet, mediante l'utilizzo di una specifica *password* di abilitazione. In particolare, questo collegamento permette l'utilizzo del prodotto denominato «Sintesi» della SOGEI, attraverso il quale è possibile accedere alle informazioni presenti sui modelli fiscali inviati fino al 2004, relativi all'anno di imposta 2003 suddivisi nelle diverse tipologie: dichiarazioni delle persone fisiche, società di persone e di capitali, IRAP, IVA e serie storiche.

in quanto lo strumento in esame risulta di valido supporto nella verifica delle analisi quantitative presentate e delle relazioni tecniche e governative, ma non può sfuggire come essi continuino a riferirsi a dichiarazioni fiscali di due anni precedenti e coincidano, sostanzialmente, con quanto comunicato al Parlamento in forma cartacea. Molto resta ancora da fare in termini di riduzione dei tempi di riproduzione dei dati desunti dalle dichiarazioni e di attività di monitoraggio del gettito che possono far acquisire al Parlamento utili indicazioni per la previsione dei futuri andamenti delle entrate tributarie per la verifica delle stime sui provvedimenti fiscali. Su tali questioni, ritenendo di interpretare il sentimento dei colleghi Questori, l'impegno che posso assumere è quello di farmi parte diligente affinché le problematiche sollevate siano affrontate nelle sedi competenti.

Quanto all'ordine del giorno G2, con il quale il senatore Eufemi chiede di individuare maggiori spazi di parcheggio a disposizione dei senatori presso l'aeroporto di Fiumicino, posso assicurare che i contatti sono già in atto da tempo con la società di di gestione dell'aeroporto stesso. Peraltro, l'oggettiva ristrettezza di aree disponibili al di fuori dei parcheggi già realizzati a pagamento rende non facile tale trattativa. In ogni caso, ricordo che i senatori in carica hanno la possibilità di parcheggiare la propria autovettura nel parcheggio multipiano presso l'aeroporto di Fiumicino a prezzo convenzionato. La richiesta in questione, ove vi sia interesse da parte dei colleghi, va inoltrata al Servizio per le competenze dei parlamentari. Il costo annuale, peraltro assolutamente competitivo, è di 619,74 euro ed è attivato dagli Uffici del Senato. La somma relativa viene poi recuperata sulle competenze mensili del senatore richiedente. con riferimento all'ordine del giorno G3 il problema ivi sollevato nasce dalla conformazione strutturale del Palazzo e dalla necessità di contenere l'inquinamento elettromagnetico. Sono questi i motivi per i quali in talune Aule di di Commissione il segnale della telefonia mobile risulta insufficiente. La questione, peraltro, ha già formato oggetto di studio da parte dell'ufficio per i lavori e i servizi tecnici che, dopo aver vagliato varie ipotesi, ha ritenuto di poter ovviare a tali inconvenienti programmando l'attività di cablaggio di palazzo Carpegna che, compatibilmente con i lavori parlamentari, potrà essere conclusa entro la prossima estate. L'ordine del giorno può quindi essere accolto dal punto di vista tecnico; occorrerà però approfondire la questione anche al fine di tener conto della posizione dei Presidenti di Commissione più direttamente interessati. Ringrazio anche il senatore Paravia, che al pari del senatore Eufemi non vedo

generale sulle problematiche connesse alla tutela delle condizioni dei giovani lavoratori e collaboratori operanti in ambito Senato. Entrando nel merito dell'ordine del giorno G1, il problema della disciplina della figura professionale del collaboratore del parlamentare è da tempo all'attenzione del collegio dei Questori, anche a causa delle ricorrenti polemiche riportate sulla stampa. Quindi, l'ordine del giorno interviene su una materia, di cui adesso dirò, della quale ci siamo già occupati. i competenti uffici dell'amministrazione del Senato sono stati invitati prima ed hanno fatto poi un approfondimento di tutta la tematica. Cosa emerge da questo approfondimento? Da una prima disamina è emersa tutta la complessità della questione: è un tema delicato al quale inviterei anche i colleghi che si sono impegnati in altre a dedicare un po' di attenzione perché questa problematica è oggetto di interlocuzioni, anche da parte di tanti cittadini nei rispettivi collegi; almeno, per me è stato così. così. Tutta la complessità della questione va affrontata sotto il triplice profilo degli aspetti fiscali, contributivi ed assicurativi nonché normativi in senso stretto. A quest'ultimo riguardo vi è l'evidente difficoltà di conciliare la natura fiduciaria del rapporto con il quadro delle figure previste dal vigente ordinamento in materia di diritto del lavoro. Da qui anche la problematicità delle risposte che il collega Paravia citava nel suo intervento, sia quelle del Ministro che quelle dell'amministrazione. Ebbene, per risolvere in modo certo ed univoco l'insieme di tali problematiche, che direttamente o in modo riflesso sono collegate alla figura professionale del collaboratore del parlamentare, appare indispensabile un intervento normativo primario *ad hoc*, cioè specificatamente dedicato a questo tipo di situazione. Quindi, spetta soprattutto all'iniziativa legislativa dei Gruppi parlamentari individuare le opportune soluzioni, che siano condivise ed allo stesso tempo rispondenti ai vigenti princìpi in materia di rapporti di lavoro. Giustamente l'ordine del giorno del senatore Paravia esprime l'esigenza di riferimenti omogenei in questa materia tra le due Camere. Non a caso, la questione dei collaboratori dei parlamentari è stata sollevata anche nel corso della recente recente discussione sul bilancio interno della Camera dei deputati, in cui è stata accolto come raccomandazione, seppure genericamente e senza l'assunzione di impegni precisi, uno specifico ordine del giorno che, peraltro, si limitava a sollecitare un ausilio di tipo amministrativo nella gestione dei versamenti diretti. Da parte nostra, non vi sono difficoltà a riferire alla prima occasione utile di un incontro con i colleghi Questori della Camera sul problema sollevato e sull'esigenza manifestata di garantire la dovuta e completa tutela dei collaboratori.

il doveroso impegno di fornire tutti gli opportuni suggerimenti tecnici, ovviamente con l'ausilio dell'Amministrazione del Senato e, se necessario, anche mediante appositi incontri con dirigenti delle amministrazioni pubbliche competenti in materia fiscale, contributiva ed assicurativa. Con questo spirito fattivo può essere accolto l'ordine del giorno del senatore Paravia, ma con la consapevolezza - devo precisarlo, per doverosa onestà intellettuale - che, per risolvere in modo chiaro e certo la questione della disciplina applicabile ai collaboratori dei singoli parlamentari, è

non solo nel Consiglio di Presidenza, ma anche nella Conferenza dei Capigruppo prima che il Consiglio di Presidenza assumesse quella determinazione che è contestata dal contenuto dell'ordine del giorno. Come è noto, entrambi gli organi - la Conferenza dei Capigruppo e il Consiglio di Presidenza - si sono espressi in favore della previsione,

sia dalla Conferenza dei Capigruppo che dal Consiglio di Presidenza, il quale, dopo, ha formalizzato l'orientamento, gli uffici hanno avviato le procedure di consultazione dei Gruppi ai fini dell'assegnazione dei posti

Infine, quanto alle considerazioni espresse dal senatore Boccia, che ringrazio per le espressioni di apprezzamento per il bilancio in discussione, non vi è dubbio che entro il prossimo febbraio, trattandosi di un anno di passaggio ad un nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, insieme al bilancio di previsione 2007 saranno discussi anche i due rendiconti, uno relativo all'esercizio finanziario 2005 e l'altro all'esercizio finanziario 2006. Esprimo parere favorevole sulla sua richiesta di istituire uno sportello unico a disposizione dei senatori nei pressi dell'Aula, e comunque a Palazzo Madama. Il parere è favorevole perché

che ulteriormente rafforza questo orientamento. Per quanto riguarda la messa a disposizione di postazioni di lavoro vicine all'Aula, si può suggerire l'utilizzo della sala Koch, che è una sala poco conosciuta, ma che dispone di circa 20 postazioni di lavoro ed è attrezzata con 22 *computer* aperti liberamente ai senatori, sui quali è possibile consultare le agenzie di stampa, navigare su Internet e redigere documenti da inviare immediatamente per posta elettronica o da copiare su chiavi USB. Vi sono inoltre cinque postazioni dello stesso tipo nella sala Maccari. Ricordo, inoltre, che per l'accoglienza degli ospiti tutti i senatori possono, su richiesta naturalmente, disporre di spazi adeguati nei pressi della portineria di piazza Madama, dove ci sono due sale a questo dedicate. Stamattina c'era una delegazione argentina che è stata accolta e ricevuta in quegli spazi. Assicuro il vice presidente Calderoli che l'annosa questione dei bagni, per la quale c'è stato un particolare impegno della collega Thaler Ausserhofer, sarà oggetto di ulteriore attenzione da parte dei senatori Questori. Aggiungo che è già allo studio degli uffici competenti un progetto di riqualificazione complessiva dei bagni situati nei pressi dell'Aula. Infine, ringrazio ancora il senatore Morando, al quale posso assicurare che le preziose riflessioni svolte nel corso del dibattito sono e saranno, per i senatori Questori, un patrimonio di utili indicazioni in ordine alla più corretta e rigorosa gestione del nostro bilancio. Assicuro anche a tutti i colleghi, ai quali va il ringraziamento mio personale e dei miei colleghi Questori, che siamo e saremo impegnati a garantire il massimo delle risorse disponibili alle esigenze di governo dei servizi - come ha chiesto il collega Morando - affinché le nostre strutture ed i senatori godano sempre di condizioni ottimali per l'espletamento delle delicate funzioni parlamentari. Una prima fase di questa situazione di emergenza, che abbiamo ereditato e trovato all'inizio della legislatura,

dopo i lavori di ristrutturazione, di nuovo fruibile per i servizi del Senato e per i colleghi. Sappiamo tuttavia che il problema che il problema della fruibilità e della utilizzabilità degli spazi potenzialmente disponibili non è finito; resta una fase di transizione che speriamo di concludere al più presto, perché ciò è la condizione assolutamente necessaria e indispensabile affinché sia garantito a tutti i colleghi, e al Senato in generale, un ordinato e proficuo

Per quanto la normativa sia criticabile - lo ha dimostrato adesso l'intervento del senatore Questore - credo che l'Aula del Senato non dovrebbe mai dire che c'è un'incertezza normativa che determina evasione fiscale e contributiva. Credo infatti che, se i senatori oggi vogliono, anche con le leggi attuali, di evasione fiscale e contributiva non ne fanno. Quindi, dire che quell'incertezza determina evasione fiscale e contributiva da parte dei senatori mi pare ampiamente discutibile.

le garanzie ai collaboratori sul piano economico, della loro tutela (sotto il profilo dei diritti e così via), ma che si chiede semplicemente che ci sia una legislazione tipo

dei Questori: ad adottare, con immediatezza e preferibilmente in modo omogeneo con l’altro ramo del Parlamento, misure concrete e idonee per la dovuta e completa tutela dei collaboratori,

soluzione, per le vie che sono necessarie, attraverso contatti diretti. Credo che la questione sia assolutamente risolvibile senza ulteriori rigidità.

il suo *unicum,* senza una serie di contaminazioni che non è il caso di continuare a perpetuare. Lo dico per inciso, perché vorrei ricordare a tutti l'impegno che avevamo assunto. Ora,

che hanno fornito non soltanto spunti interessanti ma anche chiarimenti che ritengo esaustivi, tanto da orientarmi verso un voto favorevole a questo bilancio. Sono certamente connesse con il bilancio interno del Senato problematiche di alto spessore, che qui non sono state trattate ma che sottostanno al dibattito di numeri e cifre che in questa sede si è sviluppato, riguardando l'incidenza del sistema elettorale sulla qualità e la composizione del Parlamento e sulla vitalità del suo funzionamento.

qualche tempo fa il presidente Andreotti, la centralità istituzionale che la nostra Costituzione assegna al Parlamento. Ma in questa sede è sufficiente affermare che le tematiche di tale tenore non sono dimenticate e concentrare l'attenzione, per ragioni di tempo e anche pratiche, su questioni inerenti la nostra quotidianità. Vorrei cogliere alcuni aspetti che sono stati ben puntualizzati e fare poche riflessioni su altre questioni non compiutamente toccate. Qualche tempo fa, signor Presidente, un anziano commesso mi esprimeva tutto il suo imbarazzo e rammarico per il degrado e per l'affievolimento d'immagine che ha subito anche il modo di rapportarsi del personale con i senatori della Repubblica. C'è una differenza da quando sono entrato io nel 2001 rispetto ad oggi, credo che anche altri colleghi più anziani abbiano notato questa differenza; non siamo certo a palesi mancanze di rispetto, ci mancherebbe altro, ma ad una certa sciatteria sì, il che più che offendere il senatore è allarmante e triste segnale di assenza di consapevolezza del ruolo e del luogo di chi è chiamato ad operare a qualunque titolo in questa sede. Occorre cominciare a rilevare che sul piano retributivo il Senato offre condizioni del tutto eccezionali rispetto ad altri livelli di pubblico impiego, più marcata se non eccezionale dovrebbe essere pertanto la risposta in termini, oltre che di professionalità, di tratto e di estetica comportamentale; se necessario, si attivino appositi corsi sulle modalità operative e comportamentali che un'istituzione di questo livello richiede. Quanto alla strumentazione conoscitiva di cui il nostro lavoro abbisogna, va riconosciuto che il Servizio studi e gli uffici di segreteria delle Commissioni hanno un alto livello di qualità per i supporti che forniscono; carente invece appare la disponibilità di quelli che il presidente Fanfani chiamava «colloqui integrativi del dibattito parlamentare», attraverso i quali, con il contributo di esperti, migliorare le nostre conoscenze sui temi sui quali siamo chiamati a legiferare. quindi, che abbiano più il taglio di seminari che di conferenze sull'universo mondo, più utili ad esigenze di pubbliche relazioni che non a quelle legislative dei singoli parlamentari i quali, tra l'altro, proprio perché parlamentari, sono più portati a ricercare e potenziare i punti di convergenza rinvenibili nella convivenza tra i popoli che ad enfatizzarne gli aspetti di divergenza. Stante la lontananza dall'Aula e dalle Commissioni della Biblioteca Spadolini, ho trovato molto utile la strumentazione informatica e bibliografica della sala Koch che ha ricordato il senatore Nieddu; egregio senatore, lei non ne ha fatto cenno, ma corrono voci su una sua disattivazione o comunque su limitazioni della sua fruibilità. Spero siano infondate, lei non ne ha parlato. Invito comunque il Presidente e i senatori Questori a valutare attentamente la questione: nei vari Palazzi del Senato abbondano le aule per convegni o ricevimenti e non si vede quale ragionevole motivo debba spingere a privarci di questa utilissima struttura, sempre che le voci raccolte siano fondate. Sono stato sempre attento a tutto ciò che può effettivamente migliorare l'immagine del Senato e i supporti di documentazione di cui possiamo disporre, in tal senso, non capiamo quale effettivo ritorno ci sia dalla dispendiosa partecipazione a mostre varie quando, a differenza di quanto avviene per qualunque azienda, l'immagine di un'istituzione parlamentare si collega al suo prodotto legislativo, che dipende, certo, dagli indirizzi politici, ma che in termini di linearità e pregio redazionale può essere migliorato potenziando le nostre già efficienti strutture interne. Non ho nulla contro i calendari, le cartoline, i fumetti illustrativi, gli opuscoli, i portachiavi, le penne, le gomme, le matite e quant'altro abbiamo sotto gli occhi nei nostri uffici e che la nostra libreria ci fornisce a richiesta. Ma perché non riprendere la prestigiosa tradizione del manuale parlamentare, sostituito da uno smilzo notiziario per i parlamentari, in cui non figura neppure l'anno di riferimento (quanto meno a me non è riuscito di trovarlo né all'inizio, né in mezzo, né alla fine dell'opuscolo)? E che dire del codice parlamentare, ottima iniziativa di qualche tempo addietro, che andrebbe aggiornata perché i nostri ordinamenti interni, più che in raccordi di settore, più o meno estemporanei, abbiano una trasparente sede di consultazione onnicomprensiva? Tutti reclamano un Palazzo più trasparente. E allora bisogna anche accentuare la pubblicità dei lavori e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei senatori Questori, degli organismi della giurisdizione interna, tutti organismi all'interno dei quali autorevoli colleghi svolgono attività pregevoli e proficue, di cui non si comprende perché attraverso una conoscenza adeguata non debba loro essere riconosciuto il giusto merito. Solo come titoli richiamo l'attenzione sulla fumosa normativa del rimborso forfetario delle spese forfetario delle spese di viaggio, sulla gestione delle aree di sosta, anche per le due ruote, riservate effettivamente, però, ai senatori, sul potenziamento del già ottimo servizio informatico e delle connesse tecnologie: tutto ciò per migliorare i servizi per i senatori. Mantenendoci ai suggerimenti che l'attualità propone, vorrei fare un cenno anche sullo *status* dei senatori a vita, non per commentare i comportamenti parlamentari, materia troppo delicata e ancora assai poco esplorata: resto, a diritto vigente, senatore eletto, senatore nominato, senatore di diritto sono tutti titolari di prerogative identiche. Potranno svolgersi considerazioni di opportunità, ma mai sul piano della legittimità degli orientamenti. Ciò che, però, stupisce è la differenza di *status* tra gli stessi senatori a vita, non per il fatto che tale differenza sussista (nel senso che può essere comprensibile che ad un *ex* Presidente della Repubblica si voglia riservare un riguardo diverso da quello attribuito a un senatore nominato), ma per la fonte normativa da cui tale *status* deriva. Infatti, non la Presidenza della Repubblica, non il Senato hanno definito *status* e apparato del senatore di diritto, ma la Presidenza del Consiglio, cui in via provvisoria una delibera del Consiglio di Presidenza si è in qualche modo adeguata. Non sarebbe male, dunque, che Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio e Senato, per i rispettivi aspetti di competenza (trascinamento di compiti e ruoli in ragione dell'alto ufficio ricoperto, aspetti di cerimoniale e *status* di parlamentare vero e proprio) puntualizzassero norme e rispettivi oneri - e concludo, signor Presidente - perché l'assetto complessivo dei senatori a vita - nell'ambito dei quali un cenno va fatto anche per coloro che siano stati

Mi riferisco alla novità introdotta dal prossimo anno, con la deliberazione del Consiglio di Presidenza, relativa all'eliminazione della sfasatura nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consultivo. Credo che il che il problema della continuità di bilancio costituisca una delle difficoltà che sono state sempre - non da oggi - lamentate ai fini di una consapevole valutazione, e dunque del voto, sui documenti di bilancio.

di esaminare il bilancio senza le perplessità di oggi. Oggi, appunto, ci accingiamo ad esaminare il bilancio all'inizio del terzultimo mese dell'anno di riferimento: non dico che questa sia una contraddizione in termini, ma vi sono difficoltà

discutere con cognizione di causa della gestione dei residui, insomma dei valori portanti effettivamente legati alla competenza, così come di quelli conseguenti agli interventi straordinari effettuati o a quelli preventivati nei vari anni di riferimento.

uffici, sui servizi ai senatori e più complessivamente sull'istituzione Senato, sia una questione che resta comunque aperta. Do atto volentieri al senatore Nieddu - anche da qui la motivazione

di riconsiderare eventualmente la denominazione dell'ex hotel Bologna, perché tutte le volte fa tornare alla mente i periodi dell'annosa ristrutturazione e le vicende legali.

con ricorso del 2 marzo 2006, il tribunale di Roma - Sezione I civile ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 giugno 2004, ha dichiarato che il fatto oggetto del procedimento civile pendente nei confronti del senatore Emiddio Novi concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-*ter*, n. 5/XIV Leg.). Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 18 luglio 2006, n. 320, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio. La questione se il Senato debba costituirsi in giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 21 settembre 2006. Nella seduta del 26 settembre 2006 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, a maggioranza, in senso favorevole alla costituzione in giudizio. Se l'Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la Giunta,

il Senato approva ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento civile pendente nei confronti dell'onorevole Nando Dalla Chiesa, senatore all'epoca dei fatti, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e pertanto ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 18 luglio 2006, n. 320, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio. La questione se il Senato debba costituirsi in giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 21 settembre 2006. Nella seduta del 26 settembre 2006 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, a maggioranza, in senso favorevole alla costituzione in giudizio. Se l'Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.